L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.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

L'ordine del giorno della seduta di domani, con inizio alle ore 10, prevede la deliberazione su una proposta di questione pregiudiziale, ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento, in ordine al decreto-legge proroga emergenza Covid-19, le ratifiche di accordi internazionali e la discussione del disegno di legge costituzionale, già approvato dalla Camera dei deputati, concernente l'estensione dell'elettorato per il Senato. Restano confermati, per la seduta di giovedì 10, il sindacato ispettivo e, alle ore 15, il *question time*, con la presenza dei Ministri dell'interno, della difesa e per le pari opportunità e la famiglia. L'Assemblea e le Commissioni non terranno sedute nella settimana dal 14 al 18 settembre, in occasione della tornata elettorale del 20 e 21 settembre. L'Assemblea tornerà a riunirsi mercoledì 23, alle ore 10, e giovedì 24, alle ore 9,30, per il solo esame del decreto-legge proroga emergenza Covid-19, approvato dalla Camera dei deputati, in quanto la settimana sarà prevalentemente dedicata ai lavori delle Commissioni, con particolare riguardo al decreto-legge per il sostegno e il rilancio dell'economia. **Calendario dei lavori

grazie.

del *referendum* sulla riforma costituzionale prima di affrontare un altro passaggio assolutamente importante su questo tema.

Gruppo Forza Italia è favorevole alla proposta formulata dal presidente Romeo, che ha perfettamente motivato la questione. di come la si pensi su questa proposta e su questo disegno di legge di revisione dell'elettorato del Senato, che dovrebbe essere discusso, secondo il calendario, proprio nell'ultima seduta del Senato prima delle votazioni su un *referendum* che riguarda di nuovo il Senato (perché riguarda la riduzione del numero dei parlamentari sia alla Camera sia al Senato), accavallare le due questioni confonde le idee, già abbastanza confuse: per un'informazione molto scarsa sui mezzi di informazione a proposito del *referendum*; per il fatto che i *referendum* si svolgono abbinati a importanti elezioni regionali (e questo non era mai successo in passato);

un'adeguata discussione (che peraltro, sul disegno di legge di cui stiamo parlando, quello sull'estensione dell'elettorato del Senato, sembra

ma sicuramente non nell'ultima seduta prima delle competizioni elettorali e referendarie. Certe questioni, in particolare relative alla Costituzione, bisogna esaminarle con una certa attenzione, 49 milioni di italiani che vengono chiamati a votare il 20 e 21 settembre. Indipendentemente da quello che diranno su una questione riguardante lo stesso organo, cioè il Senato - oltreché, naturalmente, la Camera - diciamo: comunque decidiate, facciamo anche un'altra cosa. Le due questioni non possono essere

costruzione che deve avere le sue ragioni e i suoi equilibri. Se vogliamo fare gli "spottini", allora si può andare avanti così. Se si vuol fare una riforma seria, bisogna agire in un altro modo. Senatore Malan, se posso riassumere, comunque la sua proposta di modifica del calendario è la medesima avanzata dal senatore Romeo.

si metta in ascolto della relatrice, che ha cominciato la sua esposizione. Cortesemente, colleghi, se abbassiamo i toni delle discussioni personali, io *in primis* ho l'opportunità di ascoltare la relatrice, grazie.

grazie.

la violenza, del suo vissuto e della sua storia. Ci sono il rispetto per lei, una capacità di ascolto e soprattutto professionalità e specializzazioni. Bene, per noi i centri antiviolenza sono sicuramente l'anello più prezioso dell'intera catena ed eccellenze senza le quali il sistema complessivo della rete oggi in Italia non potrebbe reggere. Eppure - da qui la scelta della Commissione di iniziare esattamente da questo pezzo - oggi i centri antiviolenza si mantengono, nella stragrande maggioranza dei casi,

per 6.000 euro all'anno per la loro attività. Chiedo a quest'Assemblea di capire cosa sono 6.000 euro all'anno per un'attività aperta cinque giorni a settimana,

attraverso la Convenzione di Istanbul, fino ad arrivare ai piani antiviolenza del 2014 e del 2017 e alla prima intesa Stato-Regioni, ha costruito un'impalcatura e una legislazione sicuramente di tutto rispetto. lo diciamo nella nostra relazione - è stata sicuramente la legge n. 119 del 2013, con la quale finalmente destiniamo finanziamenti strutturali ai centri e ai piani antiviolenza; riconosciamo un metodo e un approccio metodologico a questi centri, ne facciamo tesoro diciamo che quello è il metodo giusto, ma ci fermiamo lì, perché i finanziamenti sono ancora insufficienti. Soprattutto - questa è la seconda grande criticità che fotografa la relazione - non abbiamo una lettura intersettoriale e interistituzionale chiara e corretta delle relazioni tra i soggetti che operano per il contrasto alla violenza e non facciamo ancora tesoro in maniera sufficiente della lettura corretta della violenza contro le donne, che solo ed esclusivamente dentro i centri antiviolenza riesce davvero ad albergare. albergare. Lo voglio dire con chiarezza: la violenza contro le donne, per noi della Commissione d'inchiesta sul femminicidio, che seguiamo questa materia quotidianamente, è lo specchio di rapporti asimmetrici di potere che ancora esistono tra gli uomini e le donne. Non ci stancheremo mai di dirlo. Non c'entrano niente i *raptus* degli uomini, l'aggressività improvvisa di un uomo o la condizione d'instabilità e di sofferenza. Siamo stanche di leggere titoli di giornali che raccontano di improvvisi scatti di uomini alterati, che aggrediscono le donne. Non c'entra niente tutto questo. La violenza contro le donne è la fotografia di rapporti asimmetrici di potere: per questa ragione chiediamo, anche in questa sede, che sia finalmente inquadrata nella maniera corretta, quindi intersettoriale e interistituzionale, nel raccordo tra tutti i soggetti che lavorano, il che significa

Ci sono stati sicuramente interventi che hanno voluto accelerare ed aiutare in tal senso e l'impegno di tutti i governi - lo possiamo dire in maniera trasversale - è stato sicuramente volto ad accelerare i tempi, ma non ci siamo ancora. Ancora rischiamo che i soldi arrivino ai centri antiviolenza due anni dopo lo stanziamento e questo sicuramente non è un bene. lo diciamo chiaramente - che i finanziamenti siano stanziati anno per anno e non consentano programmazioni di tempo più lunghe. Chiediamo che siano almeno triennali. Non è un bene che le operatrici facciano sostanzialmente un lavoro di volontariato. Non è un bene

accelerazione, ma anche sui criteri per l'aggiudicazione delle risorse. Non è accettabile il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, non si può adottare per i centri antiviolenza. Chiediamo di superarlo e crediamo che sia un passo importante per valorizzare l'altro aspetto che appare più critico: la mancanza di specializzazione e professionalizzazione di alcuni soggetti che vengono ammessi a finanziamento. La stragrande maggioranza dei centri è fortemente specializzata, ce ne sono stati alcuni di nuova istituzione e troppe volte in questi ultimi anni si sono costruite nuove realtà per accedere ai finanziamenti senza avere quella specializzazione e quella specificità dei centri che per noi sono fondamentali e preziose. Servono criteri e accreditamenti più stringenti. Facciamo in modo di valorizzare davvero i centri che fanno di questa cultura il loro *asset* e il loro modo di operare, perché questo per noi può fare la differenza. Dal finanziamento ai centri, dalle procedure e dall'aumento delle risorse passiamo alla valorizzazione vera di questi luoghi, capendo che vi si fanno, sì, protezione e accoglienza, ma si può fare anche prevenzione, per cambiare un modo di leggere la violenza contro le donne e per farne innanzitutto una battaglia culturale, che è quella vera, che noi insieme possiamo vincere. Questa è la ragione per cui, oltre a ringraziare le tantissime audite dei centri antiviolenza e tutti gli operatori, Conferenza Stato-Regione, Dipartimento, Istat e CNR, che hanno con noi costruito questa relazione,

finestra"). Avverto che eventuali proposte di risoluzione al documento in esame potranno essere presentate entro la conclusione della discussione. Dichiaro aperta la discussione. È iscritta a parlare la senatrice Rossomando. Ne ha facoltà.

La sottolineatura allora è che questi centri hanno sicuramente l'importantissima funzione di sottrarre innanzitutto alla violenza fisica, intesa come atto concreto e minaccia all'incolumità psicofisica

perché il danno fortissimo che viene arrecato alle donne vittime di questo tipo di violenza non è ovviamente la violenza fisica in sé, ma la perdita del sé. D'altra parte, cos'è la violenza di genere, genere, se non una violenza connaturata dal voler far perdere il sé a chi ne è oggetto? Che cos'è, se non una violenza diretta all'annullamento dell'altro da sé? Che cos'è, se non la rottura di quel rapporto che non è ovviamente solo sentimentale, perché il rapporto emotivo-sentimentale con un'altra persona è il riconoscimento dell'altro da sé,

moderne. Non ci stancheremo mai di dire, infatti, che la violenza di genere e gli episodi di femminicidio sono un fatto moderno, non arcaico e il frutto di una crisi delle società moderne. Sicuramente Sicuramente non è il luogo né il momento e poi essendo cose risapute, commetterei un torto a doverle ricordare e ripetere, ma è ovvio che nel passato c'erano rapporti fermi e stereotipati di potere e di soggezione che ovviamente stabilivano una serie di criteri e di violenze interne anche alla struttura della famiglia. Oggi però si tratta di un tipo diverso di violenza, che naturalmente risente anche dell'incapacità di ripensare le relazioni tra uomo e donna. Ecco quindi, per concludere, l'importanza di ritrovare se stesse.

Sì, perché, a parte alzare la tavoletta del *water*, fare la spesa, mettere lo sporco nei cestini, badare ai bambini e poi anche partorire - perché, intendiamoci, siamo noi a dare alla luce voi uomini, e per fortuna, perché sicuramente, per il dolore che si prova, se ci fosse questa prova per voi uomini, l'estinzione dell'umanità sarebbe già un dato di fatto

amarle o che sono i loro padri. Mi rivolgo a voi uomini, perché sicuramente oggi l'esempio e soprattutto il dovere

ma in effetti è stata estesa anche alle donne e quindi sarebbe bello promuovere ancora una volta questo strumento, perché di strumenti ne abbiamo dati tanti e ne abbiamo ogni giorno perfezionati e migliorati altri. È il momento, però, di lavorare anche sulla cultura, per permettere agli uomini

il padre dei propri figli. È questo il vero motivo per cui spesso si arriva purtroppo ad acquisire il dato quando la donna non c'è più, quando viene ammazzata. Dobbiamo essere consapevoli di doverci prendere cura di chi ci ha dato la fiducia, non solo come rappresentanti politici, ma anche come donne, è il femminile che si prende cura di voi e, a parte le mie battute iniziali, ricordatevi che è la donna che è l'origine di tutto, che si prende cura di voi, della casa, dei vostri figli, degli uomini e quindi spetta a voi uomini essere da esempio e da monito per tutti gli altri affinché non ci sia questa aberrazione che è il femminicidio. Concludo invitando i colleghi ad ascoltare stasera un grande artista, il maestro Battiato, che nella canzone «La cura» afferma che che la donna è un essere speciale e che avrà cura di lei: «Io sì, avrò cura di te». È questo l'appello e la preghiera che rivolgo a tutti gli uomini: abbiate cura di noi donne perché siamo un dono da amare e proteggere. Le donne dovete conquistarle con i fatti, non solo con le belle parole, e i fiori - vi prego - lasciateli nei campi.

più ampia sulla rete di protezione che c'è oggi in Italia e sul perché sia ancora oggi necessaria una rete di protezione in Italia. Vale sempre la pena ricordarlo, perché sono numeri enormi: otto milioni di donne - sono i numeri certificati dall'Istat - su 32 milioni di donne in Italia hanno subito una qualche forma di violenza nel corso della loro vita, dalle intimidazioni alla violenza economica, alle minacce, alle percosse,

un uomo che considera la donna un proprio possesso e per questo si permette di toglierle la vita, un uomo che assume di avere una posizione preordinata e per questo si permette di picchiarla, di intimidirla, di vietarle di uscire. Sono uomini maltrattanti, molto spesso dipinti - forse per scaricare la responsabilità - come dei mostri o come delle persone dipendenti da qualche tipo di sostanza o di ossessione per il ossessione per il gioco. Invece non è così: nella maggior parte dei casi sono uomini che "funzionano" in altri aspetti della loro vita, ma nelle relazioni affettive e intime adottano questo metodo di prevaricazione, ritenendo la donna un essere subordinato e questo ha molto a che fare con il sistema culturale del nostro

cioè la potestà del marito di giudicare e di correggere la moglie in maniera unilaterale rispetto a comportamenti liberi e legittimi.

sull'aborto - per arrivare finalmente, nel 1995, ad aderire alla Dichiarazione di Pechino e ad affermare ufficialmente che l'Italia era per la parità di genere e per la valorizzazione dei talenti femminili. È solo nel 1997 che il Governo italiano ha emanato la prima direttiva contro la violenza sulle donne: parliamo di tempi recentissimi. Del 2001 il primo provvedimento precautelare per l'allontanamento di un uomo maltrattante dalla casa familiare. È intuitivo intuitivo che una donna già vittima di violenza non può subire una vittimizzazione secondaria, con l'ulteriore violenza di essere allontana insieme ai propri figli dalla casa e che debba essere invece l'uomo acclaratamente violento ad essere allontanato. Eppure, ancora oggi, c'è molta difficoltà e molta resistenza ad applicare la normativa, che solo i tempi

si concentra poi moltissimo sull'autore della violenza: non possiamo continuare giustamente ad aiutare le donne senza evitare che le donne siano vittime di violenza e per questo dobbiamo fortemente lavorare sugli uomini. l'Italia ci è arrivata, ma ci è arrivata tardi perché il primo piano straordinario contro la violenza sulle donne è del 2015-2017, per cui stiamo parlando di tempi contemporanei. Sembra quasi un'aberrazione: mentre il nostro Parlamento adottava la Convenzione di Istanbul, prevendendo un approccio integrato - quindi non solo centri antiviolenza e case rifugio, ma nuclei di valutazione con i servizi del territorio, con la polizia, con gli ospedali

mentre la Convenzione di Istanbul metteva al centro il *focus* sull'uomo maltrattante per evitare la violenza sulle donne e per proteggere la donna, noi ancora eravamo fermi

di euro, ma il costo diretto o indiretto della violenza contro le donne in Italia ammonta a 17 miliardi di euro all'anno; 17 miliardi all'anno in servizi medici, servizi sociali, avvocati. La macchina che si mette in moto è poderosa. È un'ingiustizia, ma è anche un danno enorme contro il Paese. Dobbiamo allora metterci nella predisposizione di stanziare enormi risorse per vietare che nel nostro Paese vi sia questo fenomeno, che vogliamo - forse

non ci sono condizioni economiche, sociali, di titolo di studio che differenzino questo modello di comportamento. È un modello di comportamento che prescinde, che si basa solo su una sperequazione di potere tra uomini e donne. La sfida che abbiamo davanti è allora questa, proprio nella settimana in cui iniziamo le audizioni su *recovery fund.* Usiamo le risorse del *recovery fund* per precisamente che l'Italia è dentro i principi di parità e di non discriminazione che la nostra comunità europea ci indica e a cui noi apparteniamo. Usiamo allora questi fondi per la prevenzione, per la protezione, realizzare veramente un metodo integrato di approccio alla violenza. Lo dico perché io vengo da un territorio in cui queste cose si sono già fatte. si sono già fatte. È un territorio che, potendo finanziare, con le proprie risorse, i centri antiviolenza e tutta la rete del sistema antiviolenza, può permettersi anche di guardare all'eccellenza e di porsi passi avanti rispetto al modello nazionale. Ma proprio per questo io dico che si può fare; si può fare la prevenzione, facendo i corsi di educazione al rispetto in tutte le scuole di ogni ordine e grado, in tutte le università, affinché non ci siano più giornalisti che scrivono certi titoli, non ci siano più giudici che scrivono non ci siano più medici che non riconoscono la violenza, non ci siano più Forze dell'ordine che rimandano a casa la donna dicendole di essere brava e di non far arrabbiare suo marito.

siano fatti in maniera diversa. Il metodo dei bandi annuali non aiuta la programmazione, non aiuta a strutturare servizi di qualità. Ci sono dei modelli, che ho visto nel mio territorio, di coprogettazione e di accreditamento dei centri che durano anche cinque anni, dando la possibilità di svolgere un percorso di sviluppo

Abbiamo sperimentato dei codici criptati, secretati, coperti da *privacy* che seguono la donna in tutti i suoi accessi, dal primo all'ultimo, anche se non denuncia. Adesso disponiamo di un sistema che effettua un monitoraggio solo dalle denunce in poi, ma queste sono solo il 10 per cento. Noi dobbiamo fare in modo che dal primo momento in cui una donna si approccia e dichiara di essere in una situazione di violenza ella sia, con modalità che tutelino la *privacy*, seguita accesso per accesso. Tutti questi dati devono essere raccolti, perché noi dobbiamo avere la consapevolezza dell'enormità di questo fenomeno, che mette in ginocchio il nostro Paese giorno dopo giorno. Siamo una bella squadra nella Commissione femminicidio e al Governo il ministro Bonetti è una guida per tutte noi. Abbiamo donne importanti, dal Presidente al Vice Presidente, che rispetto a questo tema

La storia del Mediterraneo e la cultura machista è esistita e ha condizionato un certo tipo di rappresentazione della donna e, soprattutto, un certo tipo di rapporto tra la donna e l'uomo:

Questo è un fondamento della nostra tradizione culturale e, quindi, è chiaro che, quando si è di fronte a un passaggio di proprietà, la proprietà

non capisci perché una tua proprietà non si comporti come ti aspetteresti. È come se uno va in cucina la notte, tenta di aprire il frigorifero per prendere l'acqua e il frigorifero si rifiuta di aprirsi; questa persona darebbe di matto.

alla mafia, che c'è un problema sul traffico e la gestione dei rifiuti, c'è un problema drammatico di femminicidio, che ovviamente è la punta dell'*iceberg* e l'elemento radicalmente più grave, ma che arriva alla fine di tanti altri aspetti di violenza e di sopraffazione. Il lavoro estremamente rigoroso fatto in questi mesi, di cui la relazione dà giustamente memoria e sulla quale però si prendono degli impegni, è collettivo. Io credo che da questo Parlamento possano uscire oggi tre messaggi veramente significativi e importanti. Vi è innanzitutto un messaggio unanime di appoggio e di supporto a tante persone, innanzitutto a chi è vittima di violenza, che deve poter sapere e che potrebbe sapere dai nostri discorsi e - ci auguriamo - da un'attenzione mediatica al tema, dai titoli dei giornali, che il clima e la cultura stanno cambiando. poi un messaggio a chi combatte la violenza, a tutti coloro che operano in questo settore nei centri antiviolenza, ma anche a tutti coloro che operano nel campo della giustizia: sappiano che il Parlamento e i cittadini italiani, che noi rappresentiamo,

stiamo facendo, ma dobbiamo fare di più perché abbiamo di fronte un'enorme sfida culturale e vinceremo e combatteremo questa piaga

la questione della violenza sulle donne è molto complessa e giustamente è stata istituita una Commissione che se ne occupa. Ringrazio pertanto il Presidente e tutti i componenti della Commissione per il lavoro che hanno svolto e per le relazioni che stanno preparando e che stanno presentando all'Assemblea, che giustamente le deve esaminare. se sembrerebbe quasi superfluo farlo, voglio dire che la violenza di un uomo su una donna è esecrabile, ripugnante e da rigettare sotto qualunque punto di vista e da qualunque versante culturale, sociale e storico la si guardi. La prerogativa della difesa della dignità della donna non è solo dell'ideologia recente, ma ogni cultura

con cui sono venuto a contatto occupandomi di altro. Presiedo da cinque anni un'associazione, che si occupa dei bambini fuori famiglia, dei bambini tolti alle famiglie, dei percorsi che devono affrontare e a volte degli abusi che vengono commessi nel togliere i bambini alle famiglie. La cosa è diventata molto di attualità lo scorso anno, quando il caso che ha coinvolto una nota località in provincia di Reggio Emilia è diventato di dominio nazionale. Il fenomeno, però, non è certo limitato solo a quell'area e non è certo nato l'anno scorso, ma va avanti da anni. Ebbene cosa c'entra questo tema con la violenza sulle donne? Alcuni casi di persone che si sono rivolte o che comunque sono

Spero di essere smentito, ma purtroppo da anni chiedo e mi informo su questa condizione e, ahimè, non

(che a volte sono vittime loro stessi, perché spesso gli uomini violenti con la loro donna lo sono anche con i bambini, e a volte no, ma sta di fatto che ovviamente ai bambini non faccia bene stare in un ambiente in cui l'uomo picchia, maltratta o esercita violenza, a volte

dal sospetto si passa all'azione. Ci sono molti provvedimenti di tribunali, che prevedono la seguente formula, riguardante i bambini di qualunque età, ovviamente minorenni: «Venga collocato il minore in uno spazio protetto

questo aspetto - «Cara madre puoi stare con tuo figlio; se però, per qualsiasi motivo, non puoi o non vuoi sia chiaro che il bambino resta qui e tu vai o dove ti pare o dove decidiamo noi».

forzosamente da queste case, perché essendo stata loro sospesa - qualche volta anche tolta - la cosiddetta responsabilità genitoriale, non hanno più alcuna possibilità, alcun diritto di stare con il bambino: hanno una facoltà di stare con il bambino. A volte, a insindacabile - di di taluni operatori, la donna viene considerata non sufficientemente collaborativa con la casa dove si trova. Essere collaborativa vuol dire naturalmente tenere in ordine la stanza o gli spazi che condivide con il figlio o i figli; ma a volte vuol dire anche fare le pulizie nelle zone comuni e le scale, non certo perché la casa famiglia abbia bisogno di questo (perché le case famiglia non badano a spese, a volte),

viene considerata non conciliante, non collaborativa, incompatibile con l'ambiente in cui si trova, e dunque viene allontanata e privata dei suoi figli. Trovo che questa sia una cosa mostruosa *(Applausi),* perché a una donna già vittima di violenza vengono anche tolti i bambini, non perché vi sia un incidente, ma con l'infamia: tu non sei degna di essere madre dei tuoi figli. E perché? A volte per buoni motivi - ci sono anche dei casi giustificati - ma a volte no. È chiaro che è un po' come l'analisi sui tamponi: più ne fai e più è facile che ci siano dei casi positivi. Lo stesso accade

Tante volte ho incontrato, parlando direttamente con le persone o con i legali che se ne occupano, anche soggetti che, privi di titoli, aiutano persone in questa situazione. Vi è un altro

debba essere allontanato il coniuge violento. È un'elementare norma di giustizia, ma spesso si dice: «Noi possiamo allontanare il marito o il compagno violento, però non siamo in grado di tenere le Forze dell'ordine davanti alla casa; violento potrebbe sempre tornare». Per cui è meglio allontanare il coniuge che subisce (che nella grande maggioranza dei casi è la donna).

Ma come, noi giustamente siamo per la piena occupazione anche delle donne quando sono in casa loro e poi, quando sono sotto la tutela diretta delle strutture pubbliche, diciamo: «Tu, donna, devi trovare un lavoro da due o tre ore perché non potrai mica pensare di fare un lavoro normale come se tu fossi un uomo»? Di queste cose bisognerebbe occuparsi, anche perché c'è un piccolo problema. Sempre sulla base di testimonianze ricevute, risulta difficilissimo capire quanto gli enti diano a questi centri che si occupano dei bambini e delle donne. Quando lo si viene a sapere, sono somme alte, assai più alte di un buon reddito. Parliamo di 100 euro al giorno, per cui madre e figlio o madre e figlia in un mese portano 6.000 euro alla struttura che li ospita. Difficilmente le spese sono superiori. Quando c'è un eccesso di compenso per un'attività c'è allora il rischio che questa attività si gonfi, travalichi e vada al di là di quello che dovrebbe fare. Siccome c'è bisogno di tutelare le persone che si trovano in queste difficoltà, di tutelare le donne e di tutelare i loro figli, quando ce ne sono, non si può fare uso sbagliato di questi soldi, perché ciò vuol dire incentivare le cattive pratiche e magari lasciare chi davvero ha bisogno senza le risorse di cui avrebbe davvero necessità.

spero sinceramente che ognuno di noi oggi in Aula abbia contezza di quello che sta accadendo in Senato. È la prima volta che la Commissione di inchiesta sul femminicidio procede ad effettuare un'indagine di monitoraggio del sistema istituzionale di finanziamento e *governance* dei servizi che operano nel campo della prevenzione e del contrasto alla violenza maschile contro le donne. In pratica, si è tentato di ricostruire il percorso delle principali tappe politiche e normative che hanno strutturato l'attuale sistema istituzionale e del ruolo primario svolto dai centri antiviolenza e dalle case famiglia. case famiglia. Ulteriore novità di questo monitoraggio è che vengono presentate e rappresentate anche alcune raccomandazioni, che possono essere utili per una complessiva riforma della *governance* dei centri antiviolenza. tra le principali criticità che sono state riscontrate dalla Commissione riguarda il sistema di rilevamento: risulta essere ormai indispensabile una revisione dell'intesa Stato-Regioni; obiettivo prioritario non più rinviabile, da intendersi come primo necessario passaggio verso l'elaborazione di una riforma organica della normativa in materia di prevenzione e contrasto ad ogni forma di violenza di genere. Vediamo, però, innanzitutto i numeri che fanno parte di questa relazione amplissima, che è, appunto, la *summa* del monitoraggio e del lavoro intenso che tutta tutta la Commissione unita ha portato avanti per lungo tempo. Le audizioni sono state tantissime, alcune emozionanti, come hanno detto le colleghe, alcune ancora più dense di numeri, proprio perché abbiamo udito tantissime associazioni per cercare di non lasciare nessuno indietro. Questa mi sembra un'operazione assolutamente innovativa, considerando che la Commissione è composta da componenti di diversi partiti. Abbiamo, però, lavorato in maniera assolutamente armonica, tant'è vero che la relazione lascia intravedere quanto il lavoro sia stato intenso e coordinato alla perfezione tra noi commissari. ai numeri. I centri antiviolenza che risultavano attivi all'atto dell'avvio dell'indagine erano 366. Di questi, ne sono stati analizzati 335, alcuni dei quali articolati, oltre che in una sede principale, principale, in uno o più sportelli diffusi sul territorio, per un totale di 647 punti di accesso. Le donne che hanno contattato almeno una volta un centro antiviolenza sono state, complessivamente, oltre 49.000. Sono 32.000, invece, quelle che hanno iniziato un percorso di uscita dalla violenza con il sostegno dei centri. Tra queste, sono 10.488 le donne inviate ai centri da altri servizi specializzati e generali presenti sul territorio e 8.711 le donne straniere. In base alla stessa rilevazione, le case rifugio operative sul territorio nazionale sono risultate essere 264. Le persone prese in carico dalle strutture di accoglienza sono state 4.483.

quantomeno una quotidianità che, purtroppo, molte volte a queste donne viene negata e anche ai loro figli. Tra le criticità riscontrate e portate in relazione vi è anche la necessaria introduzione di criteri minimi per il finanziamento dei servizi offerti, che solo in parte vengono fissati dal piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere previsto dalla legge in vigore, che si completa ora, nel 2020. In questo caso giocano un ruolo straordinario le associazioni di donne che per prime hanno inteso sopperire ad una mancanza legislativa che poi ha fatto propria l'esperienza maturata sul campo dalle associazioni. In pratica, se queste reti rappresentano oggi la risposta più coordinata e organizzata al fenomeno della violenza di genere, è proprio grazie grazie all'impegno decennale che le associazioni femminili o femministe hanno profuso su tutto il territorio nazionale. Tali associazioni, nonostante il ruolo strategico che gli viene riconosciuto, soffrono l'assenza di politiche di coordinamento e di una sostanziale valorizzazione delle competenze maturate. Ciò rende meno efficace la risposta ai bisogni delle donne che si impegnano in percorsi di uscita dalla violenza nel rispetto della loro autodeterminazione. Ad esempio, il metodo e i tempi di finanziamento dei centri e delle case rifugio è sproporzionatamente diverso da una Regione all'altra e le criticità sono tutte a discapito di una politica di coordinamento nazionale ormai assolutamente indispensabile. Questo accade nonostante sia una delle principali raccomandazioni contenute anche nel rapporto del Grevio, l'organismo indipendente del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica che è appunto formato da esperti. Le osservazioni rivolte al Governo italiano da parte del Grevio riguardano soprattutto la semplificazione e l'accelerazione dell'erogazione dei finanziamenti a centri antiviolenza e a case rifugio. In questo senso, le associazioni audite dalla Commissione hanno coralmente sollecitato un superamento di questo sistema in favore di un finanziamento diretto

Ovviamente nella relazione chiediamo che si possano rivedere le cifre regolarmente stanziate per quelli che ormai sono divenuti dei veri e propri baluardi di civiltà rispetto alla violenza di genere. In conclusione della relazione emerge con chiarezza la necessità di una programmazione centrale e di un quadro unitario di riferimento in grado di ridurre la disomogeneità territoriale, garantendo la continuità e il necessario coordinamento agli interventi e alle politiche indirizzate alla prevenzione e al contrasto della violenza contro le donne. Al fine di garantire continuità e stabilità al sistema dei servizi antiviolenza, risulta ormai indilazionabile lo sviluppo e l'implementazione di una programmazione di più ampio respiro a partire dalla necessità di finanziamenti strutturali secondo un criterio di sostenibilità per gli enti del privato specializzati. Si tratta in pratica di superare la logica degli interventi straordinari o emergenziali (è un fenomeno che non è più un'emergenza, è un fenomeno stanziale, purtroppo) e di riconoscere quindi la dimensione sistemica del fenomeno della violenza contro le donne attraverso la definizione di un impegno istituzionale di lungo periodo nel contrasto alla violenza maschile contro le donne. In pratica - e qui concludo - la Commissione della quale mi pregio di fare parte ha inteso tracciare un percorso basato concretamente sulla prevenzione e sulla formazione, che sono ormai l'unica via possibile da poter perseguire se veramente vogliamo cancellare ufficialmente dal dizionario contemporaneo la parola femminicidio. *(Applausi)*. apre una nuova finestra"). Dichiaro chiusa la discussione. Comunico che è pervenuta alla Presidenza la proposta di risoluzione n. 1, a firma di senatori rappresentanti di tutti i Gruppi parlamentari, il cui testo è in distribuzione. Ha facoltà di parlare la relatrice.

fa sue le parti finali della relazione, impegnando sostanzialmente il Governo rispetto alla direzione di marcia e ai suggerimenti contenuti nella relazione. Come ho detto nella presentazione della relazione, dopo la storia dei centri antiviolenza e dopo l'analisi delle attuali criticità,

ovviamente con dei criteri più stringenti rispetto alla specializzazione, uniti all'esperienza, per le ragioni che sono state dette da tutti quelli che sono intervenuti. Ripeto, da un lato servono risorse e dall'altro serve specializzazione. Più risorse a fronte di una maggiore specializzazione: per noi

nel Governo tutto (a partire dal presidente Conte, che è sempre stato molto disponibile rispetto all'attività e al lavoro della Commissione), sicuramente degli alleati e dei compagni di viaggio che in qualche modo renderanno attuabili le indicazioni

Signor Presidente, sono davvero grata innanzitutto al lavoro della Commissione, alla presidente senatrice Valente e a tutte e tutti e tutti i suoi componenti. Sono grata per la discussione di quest'Assemblea, che è stata sinceramente ricca di intensità e di progettualità, volto davvero di quelle istituzioni che creano la necessaria sinergia per farsi volto di una comunità, che è l'unico luogo che può restituire concretezza di speranza alle donne, troppo sole e troppo abbandonate nella tragedia di una violenza subita e troppo spesso taciuta e dimenticata. La relazione ha messo in luce alcune criticità: il tema della complessità delle procedure, della lentezza e della non certezza di un'erogazione efficiente ed effettiva dei fondi. È un dato che io stessa ho rilevato un anno fa, quando mi sono insediata come Ministro; è per questo che nel riparto allora bloccato del 2019 abbiamo voluto mettere indicazioni di di progettualità condivisa, di coprogettualità rispetto al livello nazionale, in coerenza con il piano strategico, e di monitoraggio. Tuttavia, ritengo sia importante anche lavorare su azioni di sistema. È per questo che nel riparto 2020, che è oggi all'attenzione del coordinamento tecnico delle Regioni, c'è l'intenzione di un bando e di una progettualità di alcuni fondi destinati ad azioni di sistema, perché è un sistema Paese che va costruito e rafforzato - com'è stato detto - con una molteplicità di soggetti protagonisti, nel quale certamente i centri antiviolenza e le case rifugio, a cui va la gratitudine dell'intero Paese, svolgano e debbano svolgere sempre maggiormente un ruolo nevralgico. Ciò significa formazione, sostegno delle reti territoriali, coraggio di osare temi nuovi correlati alla violenza, come la violenza economica come il tema del rapporto tra madri e figli, che è uno degli elementi oggi problematici all'interno del nostro processo. Le donne vanno infatti collocate nel divenire di una vita che va quindi resa autonoma anche rispetto alla loro autonomia finanziaria. Restituire la libertà significa anche questo e ciò va inserito all'interno di relazioni fondanti e fondative

ma soprattutto lo dobbiamo alle donne che in questi mesi ci hanno lasciato, uccise tragicamente, trucidate dalla violenza più disumana che si può immaginare: Irina, Larisa, Barbara, Bruna, Pamela, Rossella, Irma, Lorena, Gina, Viviana e Alessandra. Parliamo di un fenomeno, ma dietro quel fenomeno ci sono storie di vita, notti di silenzio lacerate, vite violentate costantemente. E lo dobbiamo a Daniela, a cui è stata

nel contrasto alla violenza contro le donne, dai centri antiviolenza alle Regioni, la Commissione femminicidio, gli enti locali, le Forze dell'ordine e tutti i componenti della cabina di regia, non solo per verificare il Piano strategico nazionale di contrasto alla violenza maschile contro le donne, ma per disegnare una nuova progettualità, eventualmente un nuovo sistema che accompagni il nostro Paese nel contrasto di questo fenomeno, ma soprattutto nella risposta alle singole vite delle donne alle quali oggi dobbiamo davvero tutto tutto il nostro impegno, sia come istituzione che come Paese.

Signor Presidente, colleghi, Ministro, questa è la prima dichiarazione di voto dopo la discussione. Oggi quest'Assemblea si deve esprimere sulla relazione relativamente alla *governance* dei servizi antiviolenza e sul finanziamento dei centri antiviolenza e delle case rifugio.

Non capita spesso che si registri piena unanimità in Commissione e molto meno frequente è che si voti all'unanimità una risoluzione in Aula. Di questo sono contenta, perché non è questa una materia sulla quale ci si possa dividere. Lo fa solo chi è miope e piccolo. piccolo. Anzi mi correggo: non è una materia, ma è una questione, qualcosa di più ampio e di più profondo, sulla quale - ripeto - non ci si può e non ci si deve dividere, a meno che non si abbia una visione miope e piccola della stessa questione. Fratelli d'Italia voterà a favore della risoluzione e lo farà perché condivide gli impegni richiesti al Governo, ma soprattutto perché condivide quanto contenuto nella relazione approvata in Commissione. Sostanzialmente, se dovessi sintetizzare, noi - e penso di poter dire noi abbiamo chiesto più risorse da impegnare nella prevenzione e nel contrasto alla violenza sulle donne, abbiamo chiesto una puntualità e una semplificazione nei finanziamenti, che sono di vitale importanza per la vita, la gestione e l'organizzazione dei centri antiviolenza e delle case rifugio. Abbiamo chiesto anche una tempistica che non fosse improvvisata, ma certa e che fosse più lunga di quella anno per anno, sapendo perfettamente che purtroppo i finanziamenti previsti ogni anno non arrivano mai a destinazione nei tempi stabiliti e che troppo spesso i centri antiviolenza e le case rifugio devono fronteggiare l'emergenza nell'emergenza, proprio perché i finanziamenti non arrivano tempo. Abbiamo introdotto altresì la parola monitoraggio per verificare l'effettiva erogazione. In sostanza un grido per diminuire, anche qui o almeno qui, i mali della burocrazia, i passaggi, i rimandi, i rinvii per l'arrivo delle risorse e anche un aggiornamento nell'intesa Stato-Regioni. In definitiva, criteri più puntuali, requisiti chiari anche per gli enti gestori. Quando si parla infatti di queste risorse, si parla di risorse che consentono nella realtà la presa in carico delle donne vittime di violenza e dei loro bambini. Non si tratta soltanto del momento emergenziale in cui si consuma per esempio la violenza domestica, ma si tratta del dopo. Ognuna di noi riceve una richiesta d'aiuto. Cosa rispondiamo quando una donna si avvicina o ci chiama e ci chiede aiuto? La dirigiamo al numero 1522, la dirigiamo ai centri antiviolenza, le diamo delle indicazioni. realtà che accolgono le donne vittime insieme ai loro figli. Stiamo parlando di qualcosa di reale, che deve essere mantenuto nella sua funzionalità e non può essere lasciato al volontariato. Esattamente come non si possono immaginare su questa materia interventi emergenziali e di segmento,

di lungo periodo e di visione ampia, oltre, molto oltre, la logica stretta dell'emergenza. Soprattutto non dobbiamo mai favorire lo scenario, che purtroppo si si crea qualche volta anche nella percezione delle vittime, che, da un lato, ci sono le Istituzioni e, dall'altro, i centri antiviolenza, cioè la realtà di accoglienza. Questa metafora, questa immagine di separazione è un paradigma che va rovesciato, ma quando purtroppo si verifica, è anche una realtà da curare e da aggiustare. Quando, per esempio, i fondi per il 2019 sono stati sbloccati nel mese di aprile, quindi ben in ritardo, il Paese si trovava in piena emergenza del *lockdown.* Faccio solo un piccolo riferimento; quei fondi sono stati sbloccati, è vero, ad aprile, ma erano già in ritardo e questo dipende dal meccanismo che purtroppo spesso diventa rimpallo di responsabilità del del riparto nella Conferenza unificata Stato-Regioni. Non può essere però materia di disputa tra Governo e Regioni se in mezzo c'è - e c'è - la vita delle donne vittime di violenza e dei loro bambini. Ora i fondi 2020

con gli uomini maltrattanti, i loro aguzzini. Dopo la fine del *lockdown* la richiesta di sostegno e domanda di aiuto è aumentata. Le strutture che abbiamo, che sono al di sotto di quelle previste e stabilite dalla Convenzione di Istanbul, non bastano ad accogliere

carattere più qualitativo - un'eccessiva diversificazione, come diceva anche il presidente Valente, nell'offerta dei servizi territoriali. Questa è una discriminazione inaccettabile,

come non possono esistere strumentalizzazioni politiche. Infatti, dobbiamo essere consapevoli che oggi noi qui diamo un piccolo contributo a una questione purtroppo metastorica e strutturale,

signor Ministro, onorevoli colleghi, il drammatico aumento del numero dei femminicidi nel nostro Paese ci dice chiaramente una cosa, servono una rivoluzione culturale in Italia e un cambio radicale di mentalità che contribuiscano a eliminare le tante - troppe - giustificazioni che vengono trovate per l'uso della violenza sulle donne.

nazionale permanente, modifiche normative affinché ci sia un canale unico di assegnazione dei fondi. Sono tutte misure estremamente opportune, proprio perché sappiamo che la situazione è drammatica e continua, purtroppo, nonostante gli interventi, ad essere preoccupante. Per giunta, la situazione è stata resa ancora peggiore

se guardiamo i dati generali propostici dall'Istat vediamo che una donna su tre in Italia ha subito una qualche forma di violenza, sette milioni di donne tra i sedici e

dunque è un fenomeno estremamente preoccupante, che spesso vede le origini di questa violenza proprio all'interno della famiglia stessa. Tra l'altro, sappiamo che è un fenomeno spesso sommerso. cento delle violenze viene denunciato, perché spesso prevale questa sintomatologia psicologica del rinunciare alle denunce a seguito di un processo di rassegnazione che si insinua. Credo, quindi, che sia un bel gesto che questa Assemblea oggi compie attraverso l'approvazione di questa risoluzione, che dà ancora più forza a quelle battaglie portate avanti, come dicevo inizialmente, dal Ministro per le pari opportunità, che sin dall'insediamento ha attivato lo sblocco di 30 milioni per quella rete di centri antiviolenza che oggi la risoluzione chiede di potenziare e che ha messo in campo anche un meccanismo di controllo per l'uso corretto di queste risorse, prevedendo progetti di microcredito per donne vittime di violenza, investendo anche risorse che questa Assemblea chiede all'unisono di aumentare: per il momento due milioni di stanziamento. stesso Ministro che ha convocato una cabina di regia proprio per la presa in carico dei diversi casi di violenza, in modo tale che anche da parte dei diversi uffici dei diversi uffici e delle diverse amministrazioni ci possa essere la messa in campo di concrete misure proprio al fianco delle donne vittime di violenza.

o anche di ricalibratura dei congedi parentali, tutte misure puntuali volte a favorire l'indipendenza anche economica della donna, la ripresa del lavoro, lavoro, per cercare di rompere quel circolo vizioso della sudditanza economica, che spesso fa sì che si creino quelle situazioni di rassegnazione e dunque di mancata denuncia e di mancata riuscita nell'emancipazione dalla violenza a cui facevo cenno poco fa. un atto che dà valore e prestigio a questo Parlamento, per il quale il Gruppo Italia Viva non può che esprimere convintamente il voto favorevole. *(Applausi)*. Signor Presidente, noi tutti ringraziamo la Commissione per questo importante lavoro che ci consegna una relazione fondamentale

mondo di matrice patriarcale, che perpetua la subordinazione e l'assoggettamento fisico e psicologico di genere fino alla schiavitù e alla morte.

spesso, all'interno di quei centri che dovrebbero accogliere con attenzione individuale le donne, si viene a perpetuare una seconda una seconda fase di discriminazione, una vittimizzazione secondaria, com'è stata definita, perché non c'è abbastanza cultura negli operatori. È necessario si faccia un lavoro per il rafforzamento di queste strutture, che sono a sostegno, ma che si incida soprattutto nella prevenzione, facendo un lavoro di accoglienza dell'uomo violento, di diffusione della conoscenza e della cultura, partendo dalle scuole, dagli operatori e anche dalle Forze Forze dell'ordine, perché altrimenti, come sempre avviene per le donne, da una violenza si passa ad altre successive che

che una Commissione lavora su questo tema in questo modo e siamo assolutamente e fermamente grati per quanto è stato portato alla luce. Per questo

Mi permetto di sottolineare un ulteriore aspetto e mi rivolgo anche al Presidente della Commissione e a tutte le componenti e i componenti, oltre che a lei, Presidente, e al ministro Bonetti.

un ruolo di indagine per cogliere costantemente i cambiamenti, l'attuazione delle nostre leggi ma anche le necessarie implementazioni, come previsto dalla Convenzione di Istanbul,

perché vi siete presi la responsabilità di fare un lavoro che serve al Parlamento, al Governo, ma soprattutto a tutto il Paese. Ciò che è emerso, e che la relazione la relazione del Presidente a mio avviso mette particolarmente in luce, è di straordinaria innovazione ed è frutto di una capacità di lettura della storia e della realtà

economico; stiamo parlando dell'economia della cura da parte di persone con specifiche competenze. Quando si parla di specifiche competenze si chiama in causa anche tutto il sistema formativo del nostro Paese: ci sono competenze

gli investimenti che devono essere fatti attraverso i progetti, nell'ambito di un ragionamento di sistema-Paese sul *recovery fund*. Noi dobbiamo sapere che questa è una parte decisiva dell'investimento sull'economia della cura, sui servizi per la cura delle persone, in questo caso, ovviamente, per le donne che subiscono violenza e per i bambini che purtroppo assistono a violenza, oltre che per

proprio il più grande investimento che questo Paese possa fare.

a maggioranza femminile, e di tutta quella rete di servizi che stanno nei territori e che la stessa proposta di risoluzione riconosce come punto di intreccio di servizi. Anche per questa ragione

Questa volta, con la risoluzione in esame su questi temi, e non solo perché stiamo parlando del dolore, della sofferenza e del superamento di un dolore - una sofferenza e una situazione strutturale

da parte del Governo. Immagino che la Commissione e il Parlamento andranno avanti su questo lavoro perché è di loro competenza. Possono essere anche promotore e promotrice ovviamente di proposte,

cambiamento e investimenti. Ce lo chiedono le donne di ogni colore politico e ogni realtà sociale perché, purtroppo, la violenza degli uomini sulle donne non si distingue tra classi classi sociali, di età e condizioni economiche. È un punto che riguarda tutta la società. Di questo dobbiamo scegliere di fare il più grande investimento del nostro Paese. L'economia della cura con il

la relazione in esame illustra gli esiti di un'indagine di monitoraggio del sistema istituzionale di finanziamento e *governance* nei centri attivi nel campo della prevenzione e contrasto alla violenza maschile contro le donne. La relazione supera la logica degli interventi straordinari ed emergenziali. Vorrebbe indicare all'Esecutivo e al Parlamento punti da cui partire per l'elaborazione di una riforma organica della normativa in materia di contrasto a ogni forma di violenza di genere.

Stando ai dati riportati, la maggioranza dei centri antiviolenza è gestita da enti privati senza fini di lucro, complessivamente 283 (pari a circa l'84 per cento per cento di questi centri sono al Nord del Paese e questo è un fatto molto grave. La Commissione, nelle sue raccomandazioni, chiede l'adozione di procedure che riducano i tempi e semplifichino l'*iter* amministrativo per l'allocazione delle risorse agli enti gestori pubblici o del privato specializzato. Purtroppo, abbiamo perso una grande opportunità con il semplificazioni, perché non ha semplificato proprio niente. E tutti sappiamo come il cancro del nostro Paese siano la burocrazia, la lentezza della burocrazia e gli infiniti passaggi nella pubblica amministrazione. L'ammodernamento di un Paese e i risparmi di una pubblica amministrazione si ottengono non con il taglio dei parlamentari, ma riammodernando la pubblica amministrazione e semplificando in modo vero la burocrazia che impasta ogni settore del nostro Paese e, addirittura, un problema La relazione raccomanda, inoltre, la modifica della normativa sulle procedure di affidamento della gestione dei servizi ricorrendo, come previsto, dal codice del settore a modelli alternativi rispetto a quello previsto dai contratti degli appalti pubblici. pubblici. In questo contesto chiediamo anche di adottare dei criteri seri per l'accreditamento dei centri.

La Commissione ha evidenziato l'assenza di un controllo preliminare all'assegnazione dei finanziamenti sull'organizzazione del privato sociale, che già gestisce o si candida a gestire i centri antiviolenza e le case rifugio. Il timore è che le risorse vengano assegnate anche a organizzazioni di scarsa esperienza, o il cui operato non promuova il rispetto dei principi fondamentali, come la parità tra uomini e donne e i diritti umani. Non voglio dilungarmi sui numeri relativi alla violenza sulle donne - cari colleghi - perché se

i fondi per poterlo fare, mette a repentaglio non solo il buon esito, ma anche la vita stessa delle donne assistite. Molti centri antiviolenza sul territorio attendono da otto anni l'accreditamento per ottenere il pagamento delle rette delle case rifugio. Ho apprezzato moltissimo le parole del Ministro e le sue promesse: capisco che conosce questo argomento molto meglio di noi, visto che è il Ministro delegato ad occuparsi di questo tema, ma magari oggi un po' più di attenzione a quanto diciamo in Assemblea sarebbe stata gradita. Occorre riconoscere il ruolo dei presidi sul territorio, che sono una rete fondamentale per salvare la vita delle donne. Anche a questo riguardo abbiamo insistito molto su quanto il fenomeno della violenza sia strutturale, multiforme, sociale e pervasivo.

tanti altri provvedimenti; sono stati stanziati 67,2 milioni di euro per il potenziamento delle case rifugio, a cui si sommano i 77,8 milioni di euro per l'attività di prevenzione e protezione del Piano di azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere 2015-2017. Nel periodo compreso tra il 2013 e il 2019, in Italia si sono stanziati 145 milioni di euro per realizzare l'azione di contrasto alla violenza contro le donne. L'analisi della Commissione, però, parla di un loro utilizzo frammentario e lento e riporta l'inadeguatezza di molte amministrazioni responsabili dell'attuazione degli interventi ad agire in maniera puntuale contro un fenomeno, che richiede una chiara volontà politica e un impegno quotidiano, di trecentosessantacinque giorni all'anno. Il rapporto Grevio - come è stato ricordato - ha sottolineato il grave ritardo per la distribuzione dei fondi e questo è - come già detto - un ostacolo alla continuità e alla qualità dei servizi. Un'altra conseguenza di siffatto modo di distribuire fondi nazionali è la mancanza di trasparenza e di uniformità nella gestione delle risorse a livello regionale e locale. Non si ha contezza di ciò - questo lo chiedo da anni e l'ho fatto anche nella Commissione di inchiesta della scorsa legislatura la relazione di oggi è un primo passo per poter sapere con esattezza a quanto ammontano i fondi destinati al contrasto alla violenza sulle donne e come vengono gestiti, perché c'è abbastanza confusione. Sebbene vi sia stato quindi un incremento progressivo dei fondi, per le case rifugio e per i centri antiviolenza, nessun miglioramento è stato registrato rispetto alla riduzione dei tempi di assegnazione e di stanziamento delle risorse. Il tempo medio di un anno, trascorso tra l'emanazione del decreto di ripartizione e il trasferimento dei fondi nelle casse regionali, impatta negativamente sulla gestione delle risorse a livello territoriale, gravando soprattutto sulla sostenibilità delle case rifugio. In questa logica, fondamentale è l'istituzione di un sistema di monitoraggio e valutazione periodica di impatto. Per quanto riguarda le Regioni, il monitoraggio fatto dalla Commissione ha evidenziato sì segnali di miglioramento rispetto allo scorso anno, ma altrettanto il permanere di una situazione critica generale. I dati mostrano un lieve incremento nella percentuale di liquidazione dei fondi del biennio 2015-2016 per il 2017 l'attivazione e il potenziamento delle case rifugio antiviolenza in Italia. Gravissimo è lo stato dell'arte per le risorse relative al 2018 e al 2019. Dai dati reperibili risulta che, per l'annualità del 2018, solo la Regione Molise ha liquidato una quota dei fondi assegnati, mentre le restanti Regioni non hanno ancora trasferito alcuna risorsa statale agli enti locali e al privato sociale che gestiscono le strutture di accoglienza. Per l'annualità del 2019, il Dipartimento delle pari opportunità ha emanato il decreto di ripartizione dei fondi solo lo scorso aprile, e conosciamo il momento che abbiamo appena vissuto. vissuto. Questa situazione mette seriamente a rischio la gestione delle case rifugio e dei centri antiviolenza, ed è urgente attivare politiche nazionali, regionali e locali fondate su un'analisi strutturata dei bisogni. Sono molto felice di quanto è stato discusso in Commissione, della relazione presentata e votata all'unanimità; altrettanto sicura sono che sarà approvata da quest'Aula, ma spero e mi fido delle parole dette dal Ministro per poter compiere dei passi avanti concreti sulle problematiche messe in evidenza dalla nostra relazione. Signor Presidente, la Commissione, a seguito di audizioni, documentazione e testimonianze, presenta oggi in Aula un atto di indirizzo, riconoscimento dell'impegno notevole e difficile degli uomini e delle donne che si prestano alla risoluzione di una problematica complessa e articolata nei centri antiviolenza e nelle case rifugio. L'incolumità e la sicurezza delle donne vittime di violenza e di abusi è motivo di vita delle Forze dell'ordine tutte, dei servizi di tutela e di tutti i volontari che accolgono, aiutano, ascoltano e proteggono le vittime di violenza. loro va il più sentito ringraziamento. Un doveroso e particolare ringraziamento lo rivolgo ai parroci che, nel silenzio, spesso sono la prima speranza di salvezza per molte donne sfortunate. La politica deve fare la propria parte; in modo particolare la Commissione d'inchiesta deve mostrare preparazione, responsabilità e libertà da preconcetti e logiche di partito. La Commissione ha redatto la risoluzione sollecitata dalle necessità e dalle richieste, più o meno celate, di oltre 350 centri antiviolenza e di oltre 250 case rifugio. Si rivendica chiarezza, già a cominciare da un numero certificato di tali strutture, e si chiede che rispettino requisiti strutturali omogenei. Non sempre, infatti, sono operative in esse figure professionali, accreditate o specializzate, come richiesto dalla Convenzione di Istanbul. La Commissione è stata informata e ha compreso che i centri misti, le cui finalità non sono solamente specifiche alla sfera della violenza sulle donne, non possono rappresentare al meglio il luogo finalizzato alla sicurezza e alla incolumità fisica e psicologica. Occorrono centri, case rifugio e strutture specializzate e preparate alla complessità del fenomeno della violenza sulle donne e di tutto il contesto che lo circonda, fino ad arrivare alle conoscenze delle diversità religiose e culturali. La risoluzione evidenzia, inoltre, la problematica della distribuzione dei fondi disponibili, non solo limitandoli attraverso la specializzazione tali centri, ma anche e soprattutto scongiurando scongiurando il dubbio che alcune strutture possano diventare un vanto e una conseguenza politica, delegittimando l'intento e la natura notevole degli stessi. Per la Commissione è un dubbio inaccettabile. Allora occorrono criteri di distribuzione economica categorici e omogenei e requisiti strutturali e professionali obbligatori per i vari centri antiviolenza; il metodo non della raccomandazione per conoscenza, quanto piuttosto della meritocrazia nel finanziare progetti e strutture. Inoltre, nella Conferenza Stato-Regioni si sono deliberati 30 milioni: 10 milioni per centri antiviolenza, non solo pubblici ma anche privati, e 10 per case rifugio, non solo pubbliche ma anche private. I fondi, senza programmazione necessaria, sono del 2019 e la Commissione la Commissione rivendica che le associazioni stesse chiedono velocità nella distribuzione economica. È fondamentale avere una certezza per programmare e garantire, con efficacia, la qualità del servizio di assistenza e di recupero. Il periodo di emergenza Covid-19 è stato testimonianza Le figure professionali specializzate sono essenziali per affrontare e gestire il fenomeno della violenza fisica e morale. Ma, oltre al coraggio e al gran cuore, per i quali non c'è cifra che ne ripagherà l'impegno, esse vanno stipendiate e riconosciute per il lavoro effettuato. Premesso che l'unico percorso per chi abusa delle donne è una pena vera e duratura, in ambito normativo si è fatto tanto, anche se mai troppo. Nel 2009, l'Italia ha introdotto già il reato per atti per atti di persecuzione; nel 2013, c'è stata la ratifica della Convenzione di Istanbul; nel 2019, la legge Codice Rosso. Le associazioni ci chiedono anche un aiuto effettivo e concreto. Il rapporto Grevio afferma che normare è più facile dell'azione programmatica di contrasto, ma questa deve iniziare già nelle famiglie e nelle scuole e passare anche per programmi mediatici, con atti di sensibilizzazione, controllo e condanna di mitomanie negative. Le regole, le richieste e le problematiche si moltiplicano quando, nelle strutture antiviolenza, oltre alle donne vittime ci sono anche i figli. insieme al vuoto assordante sulle donne e ragazze disabili vittime di violenza, dovrà essere il punto di partenza per la prossima risoluzione. Nell'ordinamento giuridico italiano, infatti, non esiste ancora una specifica normativa a loro tutela. c'è tanto da fare. Sicuramente questa risoluzione è il continuo di una serie di battaglie di contrasto alla violenza. Al Governo si chiede oggi di implementare risorse, di specializzare e indirizzare centri e strutture antiviolenza, velocizzare e ottimizzare le erogazioni di denaro, premiare e riconoscere specifiche figure professionali, controllare i progetti ed erogazione di somme del fondo disponibile. Mi permetto, signor Ministro, visto che siamo in fase di sollecitazioni, di ricordarle che manca ancora la firma sul decreto del Presidente del Consiglio in merito all'obbligo di esposizione della cartellonistica del numero verde 1522 nei locali. Penso che si possa immediatamente porre rimedio. Come Commissione di inchiesta siamo in doverosa disponibilità a partecipare fattivamente a tali impegni e chiediamo che la risoluzione venga accolta da tutti, ma a tutti chiedo di non fermarci qui. onorando e commemorando in quest'Aula, con immensa tristezza, Willy Monteiro Duarte, morto a ventuno anni: per la mamma, il suo piccolo gigante che voleva fare il cuoco; un ragazzo d'oro, che amava amare, fino a rischiare la vita per difendere un amico. Ci stringiamo con cuore e con forza alla sofferenza dei familiari. A te, Willy, la terra sia lieve.

oggi siamo chiamati a votare una risoluzione che è figlia di un lavoro corposo, tra audizioni ed approfondimenti, sulla *governance* dei servizi antiviolenza, fatta all'interno della Commissione d'inchiesta sul femminicidio nonché su ogni forma di violenza di genere che ho l'onore di presiedere, come Vice Presidente, e all'interno della quale mi occupo di prevenzione. Ebbene, al fine di espletare un'azione preventiva davvero efficace, così diffusa e capillare sul territorio nazionale già a partire dagli anni Ottanta e Novanta - all'epoca i centri antiviolenza e le case rifugio hanno dato prova dell'importanza sociale che rivestono come punti di riferimento - sarà utile attivare dei meccanismi di controllo del finanziamento, più attenti alla spesa, magari razionalizzandola e, soprattutto, snellendone le procedure di erogazione, per garantire una continuità del servizio sui territorio. Ritengo comunque opportuno precisare e ribadire la differenza che intercorre tra i centri antiviolenza - i cosiddetti CAV - e le case rifugio. I CAV sono strutture nelle quali vengono accolte in prevalenza donne minacciate di violenza, ma che comunque non escludono anche la presenza di uomini. Le case rifugio sono strutture che forniscono accoglienza a donne e a minori vittime dirette di violenza o traumatizzate da forme di violenza assistita. Esse garantiscono agli ospiti anonimato e riservatezza. Entrambe le strutture erogano i propri servizi a titolo gratuito. Voglio altresì ricordare in quest'Aula, e per chi ci sta seguendo,

ma, accanto a questa primaria funzione, ve ne si affiancano altre altrettanto importanti. Esse infatti erogano servizi di assistenza psicologica; organizzano gruppi di mutuo aiuto; forniscono assistenza legale; accompagnano le persone a fruire del segretariato sociale; danno un indispensabile supporto ai minori traumatizzati da violenza assistita, sostegno alla genitorialità ed esercitano mediazione culturale per le donne straniere. Dunque, la permanenza in queste strutture non è passiva. Per ciascun soggetto viene costruito un progetto di intervento il più possibile personalizzato e di orientamento ai servizi e alle risorse attuabili

fondi, con tempi ridotti e minimi, direttamente agli enti pubblici, essendo questi più vicini agli operatori e ai centri che forniscono servizi in azione in materia di contrasto al vergognoso fenomeno della violenza di genere. La Commissione d'inchiesta sul femminicidio, a seguito delle tante audizioni degli addetti ai lavori, ha rilevato tante criticità sulle quali sarà utile intervenire per attenuare o risolvere del tutto il problema. Ed è stato altresì indispensabile ricostruire le principali tappe politiche e normative con le quali è stato strutturato l'attuale sistema. Cito alcuni esempi: nel 1995 l'Italia aderisce alla Dichiarazione ONU, approvata dalla quarta Conferenza sulle donne svoltasi a Pechino, impegnandosi a dare esecuzione al programma di azione. Sei anni dopo sono state adottate nuove misure di contrasto alla violenza domestica grazie alla legge n. 154 del 2001. L'anno successivo, nel 1996, viene adottata la legge n. 66 sulla violenza sessuale. Nel 1998, nel Dipartimento pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri viene avviato un progetto pilota di ricerca, azione La rete nazionale dei centri antiviolenza e case rifugio contribuisce all'elaborazione della legge n. 7 del 2006, che prevede una nuova fattispecie di reato contro la violenza sulle donne, ovvero misure antistupro e *stalking*, attribuendo rilevanza anche ad altre forme di violenza come le mutilazioni come le mutilazioni genitali femminili. Nel 2006 viene istituita la linea telefonica 1522, la cui gestione viene coaffidata, attraverso un bando nazionale, alla rete «Le Onde-Onlus» di Palermo e un gruppo di ricercatori e ricercatrici «LeNove». Questa analisi ci ha permesso comunque di rilevare dei punti critici quali il parziale riconoscimento delle associazioni che gestiscono centri e case come esperte qualificate e titolate ad intervenire prioritariamente nella definizione delle politiche antiviolenza. Ciò è rappresentato proprio dall'intesa Stato-Regioni del 2014, che ha identificato i requisiti minimi per i centri antiviolenza e le case rifugio. Altra criticità è rappresentata dall'allocazione delle risorse assegnate all'attuazione del Piano antiviolenza e dalla lacunosità dei meccanismi di rilevamento dei fabbisogni effettivi delle vittime, dando luogo, in fase applicativa, a precarietà del regolare funzionamento di molti centri e di molte case rifugio che necessitano di flussi finanziari prevedibili, oltre che di finanziamenti atti alla programmazione dei propri interventi. La stessa criticità si ravvisa, inoltre, nelle raccomandazioni del rapporto del Grevio. Una certa irregolarità si rileva anche nelle attività di comunicazione e informazione, indispensabili per promuovere quel cambiamento sociale e culturale che costituisce il presupposto per scardinare la mentalità patriarcale che si manifesta sotto forma di violenza contro le donne per tante attività di prevenzione indirizzate non solo alle donne giovani ma ad un'intera società, poiché il problema della violenza sulle donne riguarda tutti e tutti dobbiamo esserne informati. Ebbene, è in questa direzione che il 31 maggio 2019 la Commissione d'inchiesta ha inteso indirizzare alcuni quesiti ai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome. autonome. Un quesito riguardava i criteri tramite i quali i centri antiviolenza e le case rifugio potessero avere accesso alle risorse loro destinate; la risposta fornita ha evidenziato tre modelli di erogazione delle risorse finanziarie trasferite alle Regioni sulla base del piano di riparto

Mi soffermo sui riscontri ottenuti non da tutte le Regioni, ma soltanto dalla mia Regione, la Sicilia, che si avvale del secondo metodo, ovvero provvede direttamente alla selezione e al finanziamento dei soggetti gestori dei centri e delle case rifugio. rifugio. La Regione Sicilia non ha fornito informazioni sui soggetti beneficiari degli avvisi pubblici emanati per l'assegnazione delle risorse, ma, da una verifica a campione su alcuni elenchi, risulta effettuare il riparto delle risorse in base all'articolo 5-*bis*, rivolgendosi direttamente ai centri e alle case rifugio. La Regione Sicilia ha ricevuto in media, per gli anni dal 2016 al 2018, fondi pari a un milione e mezzo di euro, oltre a ulteriori risorse nazionali per concessione di contributi per l'adeguamento di centri e sportelli a essi collegati. Voglio sottolineare inoltre che la Regione Sardegna e la Regione Abruzzo non hanno fatto pervenire alcuna risposta alla Commissione d'inchiesta. dicendo che l'insieme di queste gravi criticità si ripercuote sull'organizzazione e la sostenibilità del lavoro dei centri antiviolenza e delle case rifugio; pertanto è inevitabile che ricada poi sulle donne e sui minori. Alla luce dei risultati ottenuti, la Commissione d'inchiesta ritiene necessario implementare le risorse del sistema di prevenzione e contrasto alla violenza; nonché, proprio per snellire il percorso dei finanziamenti, promuovere un'analisi dei bisogni, coinvolgendo gli enti gestori (le case rifugio e i centri antiviolenza); adottare uno *standard* e dei principi guida tali da assicurare un progressivo miglioramento della qualità dei servizi offerti; istituire un osservatorio nazionale permanente che monitori e valuti l'efficacia e l'efficienza del sistema delle azioni di contrasto alla violenza contro le donne. Proprio in questo momento si parla di prevenzione e dell'importanza di introdurre nella scuola l'educazione emozionale; dotare la scuola di una grammatica dell'emozione sta a monte sta a monte proprio per scardinare il problema della violenza sulle donne. Voglio infine segnalare - mi avvio alla conclusione - che lo scorso luglio la Giunta capitolina ha approvato delle linee guida che orientano gli operatori già presenti sul territorio nella presa in carico integrata delle vittime di violenza. È un utile strumento all'interno del progetto "nessuna "nessuna si senta sola", grazie al quale finalmente i diversi operatori possono agire in sinergia tra loro a tutela delle donne vittime di violenza, un fenomeno sempre più emergente mano a mano che le donne acquistano fiducia nell'istituzione. L'esempio datoci dalla Giunta Raggi è senz'altro un esempio - a mio avviso - virtuoso, che va esteso a livello nazionale. Concludo dicendo che il MoVimento 5 Stelle esprime un voto favorevole

nella risoluzione appena votata, abbiamo l'obbligo di ricordare Luana Rainone di San Valentino Torio, provincia di Salerno...

in un giorno così significativo in cui impegniamo il Governo, per quanto di competenza, a intraprendere ogni iniziativa utile al fine di risolvere le questioni evidenziate nella risoluzione appena votata, abbiamo l'obbligo di ricordare Luana Rainone di San Valentino Torio, provincia di Salerno, accoltellata a morte ad appena trentuno anni. Il destino beffardo e la più assurda crudeltà umana hanno voluto che proprio in questi giorni si compisse un terribile e indicibile scempio: Luana è scomparsa il 23 luglio scorso ed è stata ritrovata venerdì scorso, priva di vita. Il suo corpo straziato è stato rinvenuto a Poggiomarino, avvolto come un oggetto nelle buste per la spazzatura, gettato disumanamente in un pozzo per le acque reflue. Questo è solo uno dei tanti casi di femminicidio che siamo purtroppo costretti a raccontare. Non possiamo dimenticare che i dati statistici mondiali sulla violenza sulle donne sono ancora oggi inquietanti e lasciano sbigottiti: una donna su tre subisce violenza e in Italia la situazione non è differente. Nella risoluzione approvata oggi ricordo che abbiamo chiesto di incrementare le risorse per l'intero sistema di prevenzione e contrasto alla violenza, semplificando e velocizzando il percorso dei finanziamenti. La politica ha il compito di monitorare eventuali vuoti normativi e l'impatto che le leggi hanno sui fenomeni deviati e sanguinari, come la violenza sulle donne. Su questo dobbiamo essere tutti uniti senza divisioni di sorta, senza se e senza ma. Casi come quello di Luana Rainone devono diventare solo un triste passato da commemorare come monito futuro. Non possiamo permettere che accadano fatti simili ancora una volta. Bisogna condannare fermamente ogni forma di aggressione, vessazione e maltrattamento. La storia di tutte le donne vittime di violenza ci addolora intimamente e ogni volta che veniamo a conoscenza di fatti di sangue che hanno la radice nell'odio di genere, ci rabbuia l'anima fino al profondo della nostra coscienza. Bisogna etichettare come violenza di genere tutti quei comportamenti che non tengono conto della volontà della donna e della sua libera autodeterminazione individuale. Questa piaga va affrontata a tutti i livelli, puntando sulle note tre «p»: prevenzione, protezione e punizione. Permettetemi di aggiungere anche la «c» di coraggio.

Ricordiamoci che la storia di Luana potrebbe essere la storia di una di noi, di una nostra amica, una nostra sorella, una nostra figlia. Sono vicino alla sua famiglia e a tutte le donne vittime di violenza di ogni genere. Riposa in pace Luana: non ti dimenticheremo.

sono trascorsi dieci anni dal barbaro omicidio di Angelo Vassallo, il sindaco pescatore di Pollica, nel Cilento. Ancora non vi sono un volto o un nome per l'autore del barbaro assassinio. Nove colpi di pistola - risuonarono nel silenzio di una notte di fine estate, troncando - da un lato - la vita di un uomo semplice, intelligente, dai rapporti umani senza convenevoli; un amministratore capace e lungimirante, ben voluto dai suoi concittadini e vero artefice della rinascita di un angolo meraviglioso della Campania, Pollica, con le sue marine, Acciaroli e Pioppi. lato, l'omicidio non è riuscito certamente a recidere o distruggere quanto di buono Angelo aveva realizzato. Egli ha portato il paese cilentano all'avanguardia per la qualità dell'ambiente e della vita, della lotta costante al degrado e alla speculazione edilizia; ha combattuto con convinzione lo spaccio di droga, realizzando un'idea di politica che non scende a compromessi o a patti sulla difesa del bene comune. Suo è il merito per aver reso Pollica la capitale mondiale della dieta mediterranea, diffondendo nel mondo gli studi dei coniugi Keys, rendendo il suo Comune l'emblema di un'alimentazione - la dieta mediterranea - e di uno stile di vita oggi celebrato in tutto il mondo e riconosciuto anche dall'Unesco. Difensore della legalità, simbolo di un Meridione sano e vero, che si rimbocca le maniche, capace di utilizzare per il suo sviluppo e per il motore economico le sue ricchezze naturali; un modello e uno stile di vita *slow* che tanti turisti e visitatori richiama e tanto interesse ha suscitato nel mondo. Il suo testimone è stato raccolto dai suoi amici e dai suoi concittadini che fieramente stanno portando avanti il suo sogno e la visione della sua collettività cilentana, capace di fare perno sulla tutela ambientale, nel rispetto della legalità. Il sindaco visionario e precursore aveva scritto un futuro per quei territori, fondato sulla valorizzazione delle loro bellezze naturali, sulla diffusione della dieta mediterranea e sull'appartenenza al circuito mondiale della città *slow*, un nuovo modo di vivere la vita e la quotidianità. A dieci anni dalla sua scomparsa il suo è ancora un delitto senza autori e senza mandanti. In conclusione, signor Presidente, sono e siamo vicini, come istituzione, alla famiglia e ai cittadini nel chiedere alle autorità competenti, alle Forze dell'ordine e alle autorità giudiziarie la ricerca della verità e della giustizia per Angelo Vassallo, il sindaco pescatore. Signor Presidente, colleghe senatrici, colleghi senatori, abbiamo parlato di donne e continuiamo a parlare di donne. Questa volta, però, parliamo sentendo parlare del cosiddetto *bonus* casalinghe - in realtà *bonus* non è - inserito nel decreto agosto, si sono illuse di vedere riconosciuto, anche se con un minimo corrispettivo, il faticoso lavoro di governo della casa e della famiglia che quotidianamente svolgono: un'illusione perché, in realtà, l'articolo 22 del decreto agosto parla di ben altro. Infatti, seppur spacciato erroneamente come *bonus* casalinghe, il fondo previsto altro non è che una quota destinata alla formazione delle casalinghe e a incrementare le loro opportunità culturali e l'inclusione sociale. Di fronte a tutto questo, colleghi, Presidente, resto basita e interdetta, perché è come se si dicesse che le donne casalinghe sono delle disadattate, staccate dalla vita sociale e magari anche un po' ignoranti, visto che le si vuole formare e aiutare in percorsi di inclusione. Ritengo tutto questo una vera offesa *(Applausi)* all'intelligenza dei 7 milioni e mezzo circa di donne che per motivi familiari, o per scelta, svolgono l'attività di casalinga, uno dei mestieri più difficili perché non ci sono ferie, né riconoscimenti monetari per l'attenzione che devono dedicare non solo alla famiglia, ma anche a quanto accade fuori dalle mura domestiche proprio per ben condurre il *ménage* familiare. Vediamo meglio questo articolo che sembra molto generoso nei confronti delle casalinghe, ma che in realtà con una mano dà e con due prende. Infatti, per accedere alla formazione che l'articolo prevede per le donne coinvolte, esse devono tassativamente avere l'assicurazione prevista per le casalinghe dall'articolo 7 della legge 3 dicembre 1999, n. 493; un'assicurazione che, presa singolarmente, non è sicuramente esosa, visto che ha un costo pari a 24 euro, ma che moltiplicata per 7,5 milioni - supponendo che questo sia il numero delle casalinghe in Italia dà una cifra pari a 180 milioni di euro. Se invece consideriamo quanto previsto dall'articolo 22 del cosiddetto decreto agosto per il fondo destinato alla formazione di ogni casalinga, otteniamo ben 40 centesimi In sintesi, il tanto decantato *bonus* casalingo non va ad affamare le casalinghe stesse, ma andrà a chi si occuperà della loro formazione e soprattutto all'INAIL che, con questo stratagemma, può potenzialmente mettere in cassa 180 milioni di euro. Meglio sarebbe stato prevedere un vero riconoscimento monetario per le casalinghe, considerando che molte di loro sono anche *caregiver* familiari.

grazie.